Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, rappresentanti del Governo, quanto accaduto in questi giorni è come per un film, un libro, una canzone: un buon titolo, un bel titolo, e poi una sceneggiatura debole, una storia un po' deludente, un testo non buono. L'irragionevole durata dei processi è nel nostro Paese motivo di sofferenza per la storia delle persone, siano esse imputate siano esse parte lesa, ed è motivo di preoccupazione per il Paese anche dal punto di vista economico, se si pensa a quanti investimenti non vengono fatti da aziende che non vogliono incorrere in contenziosi infiniti. Serviva più coraggio per affrontare non il sintomo, quale l'irragionevole durata del processo è, ma la malattia, e la malattia necessitava di una qualche forma attenta e puntuale di analisi delle ragioni. Malattia di struttura e di numeri, se è vero che per 10.000 abitanti nel nostro Paese sono presenti un giudice ordinario e uno onorario, contro rispettivamente i 2,5 e i 4,5 della Germania, per esempio; malattia geografica, se pensiamo che accanto a preziosi e piccoli tribunali esistono nelle nostre grandi città gironi infernali, come sanno quelli che hanno avuto modo di frequentarli; malattia di merito, che ha nomi dei quali forse occorreva trattare in quest'Aula, con la determinazione di voler davvero andare avanti. Il processo attuale corrisponde ad una logica di lentezza; forse occorrerebbe davvero riparlare dello strumento processuale. Bisognerebbe parlare dell'aumento di contenzioso nel nostro Paese, che è una sfida che il legislatore dovrebbe raccogliere anche in altri campi. Bisognerebbe parlare, ancora, dell'obbligatorietà dell'azione penale, oggi possibile perfino dopo la lettura di un giornale. Non si può offrire un processo costoso a tutti: costa come un'orchidea e l'offriamo come se fosse una margherita. Bisognerebbe parlare ancora della certezza della pena, che mi pare certa soltanto quando si tratta di carcerazione preventiva. Bisognerebbe parlare di profili di responsabilità che riguardano tutti i professionisti, forse anche quelli che hanno la responsabilità prima del processo. Si è scelto invece di non parlare di questo, ma di inserire uno strumento che creerà disparità tra i cittadini e, come ricordava ieri il senatore Rutelli, motivi di preoccupazione riguardo alla sicurezza, gli stessi che offrono irragionevoli indulti ed amnistie. Anche per gli interventi chirurgici i tempi devono essere ragionevoli vengono standardizzati. Quando in una sala operatoria si sceglie di razionalizzare i tempi di un intervento, si fa un'analisi delle risorse e si guardano i profili di competenza, ma non si dirà mai che un intervento che deve ragionevolmente durare due ore verrà interrotto dopo due ore. Tra qualche giorno, in quest'Aula, si parlerà di trattamenti palliativi. Ebbene, il medico che attua un trattamento palliativo in luogo di una cura è un cattivo medico, farà un danno ancora più grave. Non si usa il cortisone per l'eruzione cutanea se il problema è il fegato.

Signor Presidente, colleghi senatori, ho ascoltato con molta attenzione e curiosità intellettuale tutto il dibattito sul cosiddetto processo breve. Pur non essendo un esperto di problemi giuridici, non posso fare a meno di sottolineare la passione e la competenza di molti interventi dei colleghi di minoranza, che hanno avvertito e messo in guardia l'Aula, e l'intero Paese, sulle conseguenze disastrose che, con l'eventuale approvazione della legge in discussione, peseranno negativamente sulla futura gestione della giustizia in Italia. Di contro, il silenzio assordante della maggioranza, con il rifiuto di discutere e confrontarsi, mi ha allarmato, soprattutto perché i senatori della maggioranza hanno rinunciato al ruolo autonomo di legislatori. Insieme ad alcuni colleghi del Gruppo Misto voterò convintamene contro il disegno di legge, che solo in apparenza tenta di attuare l'articolo 111 della Costituzione e l'articolo 6 della Convenzione europea La convinzione dei cittadini è quella che l'interesse particolare del presidente Berlusconi - salvarsi da processi che chiunque affronta giornalmente nelle aule dei tribunali - venga mascherato da un provvedimento generale. Ma perché non si è voluto parlare chiaramente al Paese, avendo il coraggio di affrontare il problema personale con un decreto, magari monotematico-salvagente, e poi passare a confrontarsi in Parlamento sulle problematiche generali della giustizia, che certamente ha bisogno di una seria riforma per i cittadini? Mischiare l'interesse generale con il proprio particolare è il difetto fondamentale di questo provvedimento. Per cancellare un processo non si può sostanzialmente decidere di affossare e amnistiare di fatto migliaia di reati. È un delitto politico, signor Presidente, che la storia futura difficilmente cancellerà.

di giudizio, ma non prevede certo l'impunità degli eventuali colpevoli, quanto, al limite, una multa con un indennizzo all'interessato. Le raccomandazioni europee sui termini processuali vanno intese quali tendenziali, perché bisogna tener conto anche

troppo lunghi. Estinguere il processo solo perché lo Stato non è in grado di garantirne una durata ragionevole danneggia l'accusa e, magari, pure un'eventuale parte civile. Sarebbe come dire che, per eliminare l'ubriachezza, la soluzione è uccidere tutti gli ubriachi o che, per guarire gli ammalati, le cure non devono superare i tre mesi, altrimenti si passa all'eliminazione fisica.

In ogni caso la norma si tradurrebbe in una sorta di amnistia permanente e generale. In conclusione: giù la maschera; giù la maschera; abbandoniamo l'ipocrisia e convinciamoci che questo provvedimento, ammantato di interessi generali, serve al Principe per continuare indisturbato la sua politica, che tanti danni sta procurando al Paese. Io mi Io mi auguro che questo *vulnus* possa essere corretto alla Camera. Lo diciamo tutti: il Paese, oltre a vivere un momento di gravi difficoltà economiche e sociali, ha bisogno di riforme

tutti dobbiamo avere senso di responsabilità, senza pensare ad interessi di parte. Signor Presidente, non servono furbizie regolamentari, ma quest'Aula deve imboccare, con il suo sincero aiuto, una strada che ci porti ad approvare insieme - e sottolineo insieme - nuove regole ispirate a valori comuni. Al di là di questo vostro *blitz*,

Signor Presidente, colleghi senatori, l'Unione di Centro è da sempre favorevole ad approvare una legge sulla ragionevole durata dei processi. Per noi, infatti, ogni cittadino ha diritto di essere giudicato in tempi certi, in un processo che garantisca pienamente il fondamentale diritto costituzionale di difesa. In verità, però, la legge che oggi volete approvare serve poco o nulla a fissare la ragionevole durata dei processi ed approfitta di un sacrosanto principio costituzionale per fare un'amnistia. Ancora una volta in materia di giustizia - credo che siamo arrivati alla ventesima volta - state anteponendo alcuni interessi particolari all'interesse generale ad una giustizia giusta, certa ed efficiente. Ciò che state facendo è profondamente ingiusto, perché non ci si può sempre fare scudo di principi, di norme costituzionali e di convenzioni internazionali da tutti condivisi per risolvere alcune, poche, pendenze giudiziarie. nessuno di noi è così stolto da non capire che questo provvedimento tenta di risolvere i problemi giudiziari del Presidente del Consiglio e che la soluzione che avete individuato è quella di estendere l'indulto votato nella passata legislatura ai processi in corso che riguardano l'onorevole Berlusconi, ma per l'ennesima volta avete prodotto una norma incostituzionale dal fiato corto che non servirà al *Premier* e che comprometterà seriamente il regolare svolgimento di tanti, tantissimi processi. Voglio dire qui, con assoluta franchezza ed onestà, che l'onorevole Berlusconi non ha tutti i torti e che, secondo noi, vi è stato e vi è un accanimento giudiziario nei suoi confronti, anche se in misura minore rispetto a quanto da lui denunciato. Non ci pare - ad esempio - normale che, nei due mesi che ci separano dalle elezioni regionali, vengano fissate - credo - ben 24 udienze nei giudizi che lo riguardano. Né ci sembra opportuna la decisione di non rendere effettiva una recente sentenza della Corte costituzionale, solo perché il giudizio nel quale deve trovare attuazione riguarda il Capo dell'Esecutivo. Né si può sottoporre quest'ultimo ad un continuo peregrinare per tribunali e procure di tutta Italia, precludendogli la possibilità di svolgere la sua funzione di governo. Un'opposizione responsabile - secondo noi - deve farsi carico di questo problema, anche per rimuovere quel macigno che, dal 1994 ad oggi, rende spesse volte insopportabile la politica italiana, prigioniera di un rapporto *(Applausi dal Gruppo* *PdL)* controverso e conflittuale con la magistratura, e soprattutto perché una forza politica di opposizione deve pretendere che il Governo risponda delle cose che fa e soprattutto di quelle che non fa per il Paese. Noi vogliamo sgombrare il campo dal conflitto con la magistratura per costringervi a parlare dei problemi veri del Paese, di ciò che non si sta facendo - ad esempio - per le famiglie e per le piccole e medie imprese italiane. Cari colleghi, voi state ponendo una questione giusta nella sede sbagliata e con strumenti sbagliati. Non è con la ragionevole durata dei processi che si garantisce al Presidente del Consiglio di esercitare appieno il mandato elettorale. Lo strumento non è questo e, a furia di piegarlo a queste esigenze, lo avete reso inutile allo scopo per il quale è previsto, cioè garantire agli italiani una giustizia civile, penale ed amministrativa dai tempi certi. La sede propria e lo strumento corretto noi ve lo abbiamo indicato ed è la nostra proposta di legge sul legittimo impedimento in discussione alla Camera dei deputati. Quella dovete approvare, perché è in linea con le decisioni della Corte costituzionale ed è utile a garantire al Presidente del Consiglio di svolgere con serenità le funzioni di governo. Qui ci saremmo dovuti occupare d'altro e non ci è stato consentito di farlo. A quanto pare, la bocciatura del lodo Schifani, prima, e del lodo Alfano, poi, non vi ha fatto riflettere sugli errori commessi. E non voglio citare tutte quelle leggi che, nel corso degli anni, sono state approvate nel tentativo di evitare il conflitto tra il *Premier* e la magistratura, tutte censurate dalla Corte costituzionale. Se sommiamo il tempo impiegato a discutere e ad approvare queste leggi, che si sono rivelate inutili per il Presidente del Consiglio e dannose per la giustizia, ci rendiamo conto del tempo perduto; tempo che, se usato correttamente, avrebbe regalato all'Italia riforme vere e durature in materia di giustizia. State commettendo, per l'ennesima volta, lo stesso errore. Abbiamo accantonato la riforma dell'Avvocatura italiana pronta da mesi, la riforma del processo penale, il tema delle intercettazioni per fare in fretta e furia questo provvedimento. Il calendario dei lavori di Camera e Senato è interamente occupato da queste leggi sulla giustizia e per quattro mesi, considerate le regionali, non ci occuperemo di altro. Avete imposto all'agenda politica e parlamentare una tabella di marcia che non è in sintonia con i problemi e le emergenze che vive in questo momento l'Italia e tutto questo per approvare una legge che, se resta così, al pari di tante altre fatte in precedenza, non servirà a nulla. Per cortesia, fermatevi finché siete in tempo e provate a ragionare seriamente prima di prendere decisioni che non fanno bene al Paese. Ci sono tante cose che non vanno in questo testo che vi accingete a votare e che, con un po' di buon senso, potrebbero essere cambiate in meglio. Prendiamo - ad esempio - le modifiche che avete introdotto alla legge Pinto. Così come le volete fare, si rischia, da un lato, di esporre il magro bilancio della giustizia ad un salasso economico di proporzioni eccezionali, considerato che lo Stato si troverà, per effetto di questa legge, a dover indennizzare i cittadini per oltre due milioni e mezzo di processi civili eccessivamente lunghi, per circa 600.000 giudizi amministrativi e 38.000 giudizi contabili e, dall'altro lato, di allungare i giudizi per l'equo indennizzo di almeno un anno, con l'effetto paradossale e - se vogliamo anche un po' macabro -di rendere irragionevolmente lungo il processo sulla irragionevole durata del processo. Su questo argomento siamo riusciti solo a farvi eliminare la norma che cancellava la risarcibilità del danno non patrimoniale subito per la lentezza del processo. E che dire poi della cancellazione dei processi contabili, sorprendentemente introdotta dal relatore di maggioranza in Aula? Un vero e proprio colpo di spugna che non solo consentirà a tanti amministratori locali che hanno sperperato i soldi dei contribuenti di farla franca, ma - come ha già detto il collega Lusi - renderà inutile la celebrazione dei processi davanti alla Corte dei conti. Colleghi della Lega, vi accingete a votare una legge che mette la parola fine alla vera attuazione del federalismo fiscale: una pietra tombale sull'indispensabile controllo dei conti pubblici e degli amministratori che li governano. Da un lato, vi riempite la bocca di slogan sul federalismo fiscale, su come sarà bello vedere i cittadini che controllano i propri amministratori impedendo loro di spendere inutilmente i soldi dei contribuenti. Ma che cosa succederà quando i cittadini denunceranno gli amministratori che sperperano il pubblico denaro e i magistrati, chiamati dalla Costituzione e dalle leggi a perseguirli per far restituire loro i soldi mal spesi, non saranno nelle condizioni di farlo a causa della legge che vi state approvando? La verità è che a voi non frega proprio nulla né del federalismo fiscale né della qualità della spesa; a voi leghisti interessa solo gestire il potere locale e i soldi che vi arrivano senza alcun controllo e senza dover dare conto a nessuno. Predicate bene - poche volte, per la verità - e razzolate malissimo, tanto da esservi fatti anche voi - mica siete fessi! - una norma *ad personam* per salvare qualcuno dei vostri dalle grinfie della Corte dei conti. Complimenti per la coerenza e per la lealtà nei confronti dei vostri elettori. sono state eliminate talune disposizioni palesemente incostituzionali, sono stati rimodulati meglio i tempi cosiddetti ragionevoli di durata dei giudizi penali e, soprattutto, è stata eliminata quella norma folle e razzista che consentiva ad un truffatore, ad un corruttore o a chi commetteva un falso in bilancio, di godere del privilegio del processo breve (il più delle volte facendola franca), mentre l'immigrato clandestino poteva essere processato a tempo indeterminato. Ma restano in piedi ancora una serie di incongruenze e di evidenti storture quali, ad esempio, quelle che non tengono conto nella fissazione della durata del processo della complessità dello stesso sotto il profilo probatorio e delle parti. A questo riguardo voglio ringraziare gli amici e colleghi della Lega per aver ricordato il caso dell'onorevole Mannino che ha dovuto penare ben 17 anni per veder riconosciuta definitivamente la sua totale estraneità ai fatti di un processo. Voglio dire però alla Lega che ci fa piacere che, dopo aver insultato Mannino e i tanti democristiani onesti che si sono fatti

in giro per l'Italia, tentando di sfruttare a fini politici ed elettorali le vicende giudiziarie di tante, tantissime, persone perbene, come Mannino, avete raccontato ai vostri elettori un sacco di frottole e di bugie. Ma le citazioni quando vi convengono non bastano:

Signor Presidente, l'Italia dei Valori annuncia un deciso no a questa sciagurata legge. Senatori della maggioranza, rappresentanti del Governo: corruttori e corrotti, malversatori, autori di violenza o minaccia a pubblici ufficiali, autori di turbative d'asta, calunniatori, favoreggiatori, istigatori, contraffattori e diffusori di sostanze nocive, falsificatori, sequestratori, omicidi, violentatori, intercettatori abusivi di conversazioni telefoniche, ladri, ladri in appartamento, truffatori e ricettatori vi ringraziano. Alcune decine di migliaia di delinquenti, anche recidivi e socialmente pericolosi, vengono graziati. Viene cancellato il processo, viene cancellato il reato e potranno tornare all'opera. Oltre e molto di più di un indulto. Con l'indulto si cancellava una parte della pena ad un condannato definitivo; con l'estinzione del processo si cancella il processo, si cancellano le condanne non definitive, anche se giunte in Cassazione, anche se il giudice è nel momento di emettere la sentenza. È un'amnistia per reati puniti con la pena sino a 10 anni. Mai accaduta una cosa del genere! Decine di migliaia di vittime vengono beffate dallo Stato. Dopo aver cercato giustizia per anni, le vittime avranno dallo Stato la porta sbattuta in faccia. Aiuterete invece i delinquenti, aiuterete coloro che rendono insicuro il nostro Paese, aiuterete coloro che hanno commesso torti a tante vittime. Dite di fare ciò nel nome della civiltà e nel rispetto di tempi certi del processo penale. Le vostre cattive coscienze hanno un disperato bisogno di un alibi per ingannare voi stessi e i cittadini. Grazie, vi siete rifiutati di considerare tutte le nostre proposte di legge che dormono in Commissione. Avete detto no a tutti gli emendamenti necessari per contenere l'affanno della giustizia. Voi non volete migliorare la giustizia, non avete questo interesse, non vi interessa la giustizia. Invocate l'Europa e fate una legge che l'Europa non conosce. Voi volete la morte di 100.000 processi per salvare Silvio Berlusconi dai suoi processi e affrancarlo dalle sue responsabilità criminose. Voi stupirete l'Europa e il mondo. Per fare ciò farete un danno enorme al Paese e ai cittadini. Fate pagare un costo senza precedenti; fate una norma che non esiste in nessuna parte del mondo. Applicate ai processi in corso una tempistica che incide sull'attività processuale già esaurita, norma processuale retroattiva per fatti non da compiere ma per fatti già compiuti. L'Italia, detta culla del diritto, rinnega il diritto, rinnega princìpi millenari, diventa un Paese con leggi, nell'accezione storica, barbare. Vi siete chiesti la ragione per cui il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense, le Camere penali e l'Associazione nazionale magistrati sono contro questa legge? È questa la settima legge *ad personam*. Dopo la limitazione delle rogatorie internazionali, la depenalizzazione del falso in bilancio, il legittimo sospetto, il dimezzamento dei termini di prescrizione del reato, il lodo Schifani e il lodo Alfano, ecco la settima legge per salvare un accusato di gravi ed infamanti delitti. Su di essi si erge però il più grave dei delitti, quello di sottomettere le istituzioni ai propri interessi, con il Parlamento smarrito ed asservito. Ci disgusta l'insensibilità alla morale, all'etica, alla giustizia. Avete smarrito l'idea del bene comune e non sapete più cosa significhi l'interesse collettivo e il buon governo per il Paese. La vostra visione crepuscolare dei diritti si accompagna al decadimento della morale, alla sovversione dei valori, alla protezione del male. Arriverà la fine del crepuscolo e l'Italia e gli italiani si vergogneranno di questa deriva nefasta. Il mondo guarderà e leggerà le leggi del nostro Paese e capirà come la democrazia possa essere ridotta ad un involucro, svuotata dal suo interno. Vi assumete la responsabilità e la paternità del tarlo della democrazia, del diritto, della giustizia. Molti di voi della maggioranza lo confidano: hanno consapevolezza che questa è la peggiore legge che si potesse fare. Molti di voi della maggioranza, e lo confidano, dicono che fra qualche mese bisognerà cancellare questa legge. Non si recupererà, però, l'immenso danno provocato. E farete anche finta di indignarvi per le nostre accuse e rivendicherete la bestemmia della pretesa profondità garantista delle vostre leggi. Alzerete i toni, strepiterete, ma solo per trovare l'alibi di cui avete bisogno. Ma sarà solo arroganza, ubriacatura di potere e basso impero. Forse un giorno, ma in ritardo, chiederete scusa ai cittadini. Nella storia sarete una parentesi, simbolo del degrado, dell'asservimento ad una oligarchia e della democrazia ferita. Ieri, in quest'Aula, mentre si citava il gravissimo fatto del programmato attentato distruttivo ordito contro alcuni magistrati che combattono la mafia, una parte di quest'Assemblea ha irriso all'evocazione dei nomi delle possibili vittime. Ho provato vergogna. Sapevamo dei mafiosi che brindarono alla morte di Giovanni Falcone. *(Applausi della felicità dei mafiosi in carcere e del boato di giubilo quando la radio diffuse la notizia della morte di Giovanni Falcone e poi di Paolo Borsellino. Eravamo a questo. Eravamo a questa torbida conoscenza. Oggi abbiamo qualcosa di altro: una parte dell'Aula del Senato, ieri, ha fatto un coretto di irrisione alla pronuncia del nome di Antonio Ingroia, di un magistrato che la mafia vuole uccidere

L'Italia dei Valori continuerà la sua battaglia a fianco degli italiani onesti, con i mezzi della sana democrazia, nel Parlamento e nel Paese, contro i ladri del diritto, della giustizia, dell'uguaglianza, della Costituzione, nel ricordo dei Padri costituenti e dei servitori dello Stato caduti per la legge. *(Applausi dai

mi sembra corretto partire dalla genesi di questo provvedimento per spiegare al meglio la nostra posizione. Dall'inizio della legislatura la nostra maggioranza è intervenuta in diversi settori che si collegano al mondo della giustizia, con l'intenzione di affrontarli tutti coerentemente con il progetto di riforma generale dello Stato che vogliamo realizzare. Abbiamo già approvato la riforma del processo civile, nuove norme antimafia, nuove norme contro la criminalità e l'immigrazione clandestina; abbiamo affrontato al Senato la riforma della professione forense; il Governo, con il ministro Alfano, ha già annunciato un nuovo piano carceri ed è in discussione il grande tema della riforma della giustizia. In linea con questo percorso riformatore i nostri alleati del PdL ci hanno proposto di intervenire con questo disegno di legge sul codice di procedura penale per introdurre il principio di ragionevole durata del processo. Noi l'abbiamo valutato; abbiamo visto anche che il contenuto era del tutto simile a proposte di legge presentate negli anni da diversi autorevoli parlamentari di centrosinistra e lo abbiamo dunque sottoscritto e sostenuto prima in Commissione e poi in Aula. La necessità di garantire un giusto processo è, dal nostro punto di vista, assolutamente condivisibile. Il nostro è il Paese dei processi troppo lunghi, i più lunghi d'Europa: processi che si sa quando iniziano, ma non quando quando finiscono; processi che, invece di garantire giustizia, molto spesso creano ingiustizia, soprattutto per quei cittadini che rischiano di attendere invano, per anni e anni, una risposta da parte dello Stato. Sapevamo che questa proposta avrebbe incontrato l'ostilità da parte di molti settori della magistratura, e questo era facilmente prevedibile. La casta dei magistrati, che poi in molti casi è responsabile del malfunzionamento della giustizia, da anni che cerca in tutti i modi di bloccare leggi di riforma del settore. Si lamentano che le cose non vanno, per poi bocciare qualsiasi proposta di cambiamento. Niente di nuovo, dunque, anzi semmai la prova che si andava nella giusta direzione. Quello che non ci aspettavamo, invece, è stato il cambio di linea delle opposizioni, visto che questa legge - come ricordavo prima - ricalca diverse proposte già presentate dai responsabili per la giustizia del Partito Democratico. Cari colleghi, su questo è giusto essere chiari. Fino a pochi mesi fa, eravate favorevoli a questa riforma; poi, quando vi siete accorti che interessava uno dei tanti processi del Presidente del Consiglio, allora avete di colpo cambiato idea e avete rinnegato (questa è la parola giusta, lo ricordava ieri anche il senatore Mazzatorta) le vostre proposte. Evidentemente, questa legge per il Partito Democratico è giusta e condivisibile, se riguarda i cittadini di questo Paese; non va bene se fra questi c'è anche il presidente Berlusconi. *(Applausi dai siete voi, dunque, che avete cambiato idea, che vi siete contraddetti, che avete cambiato linea, e da questo punto di vista, dato che ci accusate di questo, siete voi che vi dovreste vergognare. E qualcuno, anche al vostro interno, ve lo ha fatto capire ieri molto chiaramente: in più occasioni, su richiesta di voto segreto da parte dei rappresentanti del centrosinistra, diversi senatori dell'opposizione hanno votato contro gli emendamenti presentati dai propri Gruppi. Senatori del PD o dell'Italia dei valori hanno votato con noi, dando ragione alle nostre proposte e dando così uno schiaffo morale a Bersani e a Di Pietro, che proprio ieri sui giornali chiedevano il massimo ostruzionismo e la massima contrapposizione a questo provvedimento. Evidentemente, il voto segreto è servito a qualcuno per rivendicare la propria coerenza *(Applausi dal Gruppo* *LNP)*. Credo che in democrazia ogni Gruppo sia libero comunque di fare quello che crede, anche di cambiare idea: questo è sicuramente legittimo. Mi permetto però di far presente che è dall'inizio della legislatura che dedicate la maggior parte del vostro tempo ad attaccare le nostre proposte, il nostro Governo, contestando e criticando tutto, dimenticandovi però che i cittadini guardano i fatti e ragionano con la propria testa. Faccio un esempio. Parlate spesso di questione morale, in nome della quale avete chiesto in più occasioni le dimissioni di vari rappresentanti del Governo.

E lo dico non solo ai rappresentanti del Partito Democratico, ma anche a quelli dell'Italia dei Valori, che sono sempre i primi a fare la morale agli altri. *(Applausi dai Gruppi* *LNP e PdL)*. cosa fate ancora con i vostri consiglieri in queste maggioranze? Perché sostenete ancora queste amministrazioni? La risposta è molto chiara: solo per garantirvi i posti di potere. Questa è la realtà! Belisario)*. Non voglio dire che non è giusto parlare di moralizzazione della politica; anzi, dal mio punto di vista, è

Perdete credibilità anche quando, cari colleghi, ci attaccate negando l'evidenza. Non potete continuare a dire che il nostro Governo non ha fatto nulla per risolvere i problemi dei cittadini.

Abbiamo bloccato il flusso dei clandestini sulle nostre coste, abbiamo affrontato la crisi economica

milioni, miliardi di euro per coprire i fondi per gli ammortizzatori sociali, che sono serviti a evitare migliaia di licenziamenti. Tutto questo lo abbiamo fatto ‑ è giusto ricordare anche questo - senza aumentare di un euro le tasse ai cittadini. La realtà è questa: nasconderla, travisarla e addirittura negarla per voi è solo controproducente. milioni di voti che avete perso alle elezioni europee e il calo continuo nei sondaggi ne sono una prova evidente. Raccontare balle non vi serve a niente, vi fa solo perdere consensi. Molti giornalisti parlamentari ci fanno presente che per noi della Lega questa è la situazione ideale: il vostro modo di fare opposizione vi divide e vi fa perdere voti, il nostro modo di stare al Governo ci fa crescere nei consensi.

Questa sarà l'occasione per affrontare assieme, se lo vorrete, maggioranza e opposizioni, le grandi riforme costituzionali che da troppo tempo i cittadini ci chiedono. Noi non le vogliamo fare da soli e siamo consapevoli, come più volte ci ha ricordato anche il presidente Napolitano, che il modo migliore per farle è in maniera condivisa e con l'apporto di tutti. Proviamo allora seriamente, una volta per tutte, a lavorare nell'esclusivo interesse dei cittadini per modernizzare lo Stato, allo scopo di migliorare i servizi e la qualità e la qualità della vita dei cittadini che vivono sul nostro territorio. Per fare questo bisogna sempre lasciare aperta la porta del dialogo, e noi coerentemente lo faremo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, approvate con questo il diciannovesimo provvedimento dell'era berlusconiana destinato ad incidere su un procedimento penale a carico del*Premier*. Questo significa più cose: che per 19 volte avete usato il Parlamento, occupandone il tempo e risorse pubbliche destinate a leggi generali nell'interesse del Paese, per fini particolari; che nonostante i vostri sforzi e gli sforzi degli avvocati del *Premier* non siete stati capaci di trovare una soluzione; che la vostra priorità è stata, di Governo in Governo, innanzitutto l'interesse privato; che non avete avuto timore a questo fine di devastare l'ordinamento creando pubblico danno; che non avete mai avuto senso di vergogna. *(Applausi dal Gruppo* Non siete stati capaci di dimostrare - è inutile che ci giriate intorno - che questo provvedimento non avrà effetti negativi decretando la fine di migliaia di procedimenti penali e, quindi, denegata giustizia a migliaia di cittadini italiani. Penso anche soltanto ai processi per colpe mediche, che richiedono normalmente un'istruttoria molto lunga e complessa. E penso, quindi, a quelle parti offese, genitori, coniugi, figli di coloro i quali per imperizia grave di un medico sono rimasti uccisi. Quando, nel precedente Governo Berlusconi, con la cosiddetta legge Cirielli avete praticamente dimezzato i tempi di prescrizione del reato, al punto che lo stesso proponente, l'onorevole Cirielli, di Alleanza Nazionale, si dimise dall'incarico di relatore perché - come egli disse - non tollerava che quella legge portasse il suo nome, suo nome, le prescrizioni (lo ha ricordato il senatore D'Ambrosio) schizzarono da 200.000 a 850.000. Ora queste cifre, già impressionanti, sono destinate ad aumentare. Non basta, perché nessun imputato avrà più interesse a chiedere riti alternativi, quindi riti abbreviati di definizione del processo: ogni difensore cercherà in tutti i modi di allungare i tempi del processo,

Il risultato, dunque, non sarà soltanto l'inevitabile prescrizione, ma anche un ulteriore intasamento della giustizia penale, anche in uffici giudiziari virtuosi, come il tribunale di Torino, come i dirigenti di quell'ufficio hanno evidenziato in Commissione. Voi affermate che lo fate per assicurare la ragionevole durata del processo, oggi intollerabile. Ma è fuori da ogni logica: è come fissare su un orario ferroviario in un'ora il tempo di percorrenza di una tratta, ben sapendo che la vecchia locomotiva che percorrerà quel binario non potrà arrivare a destinazione che in tre ore. Siamo allora venuti incontro alle esigenze di celerità del processo penale e abbiamo presentato emendamenti di merito per la sua accelerazione, ma li avete bocciati tutti, perché l'idea che vi sostiene è - a quanto pare - "tanto peggio, tanto meglio". A noi, invece, la celerità del processo pare una questione centrale e per questo vi abbiamo chiesto di discutere ed approvare i nostri emendamenti, ma senza esito. Appunto, ci sarebbe da dire: da una giustizia lenta ad una giustizia negata. Non avendo argomenti convincenti, siete passati ad altro (lo faceva ancora il presidente Bricolo): ci avete accusato di essere ipocriti e insinceri perché in precedenti legislature avevamo presentato proposte analoghe. Ora, a parte il fatto che ciò è avvenuto in precedenti legislature - appunto - non in questa - appunto - a dimostrazione del fatto che solo i cretini non cambiano idea

non conduceva alla morte precoce del processo, ma addirittura ne allungava troppo i tempi. Per non essere accusata di strumentalità e di spirito basterebbe che voi tornaste a rileggere (è a disposizione di tutti i colleghi) i verbali della Commissione Pisapia, la quale, con riferimento alla proposta Fassone e alla proposta Brutti, concluso sottolineando che a tali proposte non si può aderire «in quanto, sommando i tempi della prescrizione del reato», perché noi abrogavamo la cosiddetta legge Cirielli, «ai vari intervalli che compongono il termine temporale per la prescrizione del processo

Se studiaste un po' di più invece di incaponirvi soltanto a fare strumentalità politica, probabilmente ne guadagnerebbe anche il dibattito in questo Parlamento. Ma non vi siete fermati al processo penale. Come molti colleghi in quest'Aula hanno spiegato (da ultimo il collega D'Alia), avete rivolto la vostra puntuta attenzione anche al processo contabile. A fronte dei continui richiami, in particolare da parte della Lega, al principio di responsabilità di funzionari ed amministratori pubblici, avete così giubilato centinaia e centinaia di processi contabili, con il risultato di danneggiare irrimediabilmente le casse dello Stato ed introdurre principi di irresponsabilità per chi dissipa risorse pubbliche. Noi siamo gli stessi che insorsero contro il cosiddetto provvedimento salva-ladri dei primi anni '90 e voi, colleghi della Lega e di Alleanza Nazionale, chi siete? Chi siete più? Quanti silenzi e quanta smemoratezza ci sono tra voi! C'è un profilo politico che non può sfuggire in questa discussione se non si vuole essere omissivi: tutto questo avviene nel momento in cui - così almeno pare tornano fragilmente a mostrarsi le condizioni per una riforma costituzionale condivisa a larga maggioranza. Potremmo trarne due osservazioni: da una parte dite di essere interessati al processo riformatore, dall'altra mostrate atteggiamenti disarmanti, continuando ad avvelenare i pozzi. Eppure su di voi, Governo e maggioranza, grava la responsabilità del clima politico: da una parte vi mostrate interessati al processo riformatore, dall'altra tentate di spacciare questa come riforma della giustizia. Vedete, noi crediamo sia necessario riformare le nostre istituzioni per rendere il sistema democratico più forte e affidabile, contro i rischi del populismo e del travolgimento dell'equilibrio tra i poteri, per l'affermazione della centralità costituzionale del Parlamento e il ripristino del principio di rappresentanza. Per questa opera qui ci troverete: ma non per altro, e certamente non per questo.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, perché arriviamo all'approvazione di un disegno di legge contro l'irragionevole durata dei processi? Perché nel 1999, quando voi eravate in maggioranza, si introdusse, all'articolo 111 della Costituzione, il principio del giusto processo. Dice la Costituzione «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato della legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». L'articolo 6 della Convenzione europea

introduceva il principio del risarcimento per chi viene danneggiato da una irragionevole durata dei processi. La lentezza della giustizia è considerata da tutti, anche nelle solenni inaugurazioni dell'anno giudiziario presso la Cassazione, anno dopo anno, una delle cause principali della crisi della giustizia. Vogliamo evitare anche conseguenze onerose per le casse dello Stato: dal 2005 al 2009 sono stati versati 267 milioni di euro ai cittadini che hanno ottenuto un risarcimento per l'eccessiva durata dei processi. Diceva prima la presidente Finocchiaro che solo i cretini non cambiano idea. Allora, alcuni che non hanno cambiato idea a sinistra sono cretini, gli altri sono incoerenti: *tertium non datur* evidentemente. Molto più generose del provvedimento in discussione oggi sono state le proposte di Fassone, Maritati e della stessa Finocchiaro, che nelle precedenti legislature la sinistra ha presentato per garantire per tutti i giudizi termini più brevi che avrebbero cancellato - quelle leggi sì, ove fossero state approvate - centinaia di migliaia di processi! Non furono approvate, ed è stato un bene per la Repubblica e per la giustizia. Allora, c'è ipocrisia. Voi credevate che qualcuno si dimenticasse delle vostre proposte. Ne avete dovuto parlare perché sapete che noi non ce ne dimentichiamo e vi richiamiamo ad una maggiore coerenza e al rispetto dei principi europei e della nostra Costituzione. Non arriviamo a questo provvedimento sulla giustizia senza avere fatto prima altre cose: non siamo partiti dalla giusta durata del processo, anche se avremmo potuto farlo. Abbiamo varato la riforma del processo civile e norme severe antimafia; abbiamo inasprito il carcere duro; abbiamo avviato la riforma dell'avvocatura, che è pronta per l'approvazione; il Governo ha presentato il disegno di legge di riforma del processo penale. Siamo pronti alla riforma costituzionale sulla giustizia, che ci auguriamo condivisa, ma siete voi che dovete fare uno sforzo di coerenza ricordandovi dei principi costituzionali che anche voi avete votato perché diventassero garanzia per tutti i cittadini.

euro. Questa è la nostra politica della giustizia e della sicurezza, che noi mettiamo tutta insieme per la certezza della pena e la trasparenza della giustizia. Siamo orgogliosi di votare anche questa legge, che è un tassello di una politica importante per il nostro Paese. Vogliamo anche chiederci: ma è davvero breve questo processo? Nella legge la dizione «processo breve» non c'è: questa è la legge contro l'irragionevole durata dei processi. È una legge coerente con le esigenze investigative. Poi, se andiamo a vedere, cari colleghi, dal 2004 al 2008 in Italia processi per prescrizione dei reati; senza questa legge, che noi ci auguriamo imporrà alla magistratura di celebrare i processi, anche questa sera, prima che scocchi la mezzanotte, altri 470 processi

Quindi, è una legge che poniamo a garanzia degli onesti ed a monito dei colpevoli, per evitare che la prescrizione dei reati cancelli migliaia di procedimenti. La legge che proponiamo non cancellerà i processi. Il ministro Alfano è venuto in Parlamento con dati attendibili a dimostrare che l'impatto di questa legge riguarda l'uno per cento dei 3,5 milioni di processi in essere. Le vostre proposte, senatrice Finocchiaro, avrebbero, quelle sì, fatto strage di processi. Il ministro Alfano è venuto con dei dati attendibili in Parlamento, mentre abbiamo visto dei togati, che sembravano degli astrologi o delle chiromanti, dare numeri falsi per avvelenare un dibattito che noi portiamo avanti con coerenza e rigore. Inoltre, le norme transitorie tengono conto dell'indulto e quindi dei processi che potrebbero essere vanificati dall'applicazione delle norme sull'indulto che il Parlamento ha approvato. ministro Alfano, il Governo, tutti noi, abbiamo affermato delle verità. La Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che il tempo di un processo dovrebbe essere tra i sei e gli otto anni. La legge che stiamo approvando prevede per i reati per i quali è prevista una un tempo di sei anni e mezzo per i giudizi; se aggiungiamo il tempo delle indagini (mediamente due anni) e un eventuale ulteriore giudizio disposto dalla Cassazione

con facoltà del magistrato di allungare i tempi. Mi chiedo io: è questo un processo breve? Noi vorremmo che il prossimo Totò Riina l'ergastolo lo avesse in 15 mesi, non in 15 anni come le leggi oggi ci costringono a fare. *(Applausi

Non serviva e non c'è stato un decreto, che non sarebbe stato *ad personam,* per attuare la sentenza della Corte, che era effettiva, come dice anche Capotosti e tanta parte della dottrina.

*(PdL)*. Questa è la verità: certezza della pena, un orizzonte più sereno per chi, innocente, ha diritto a vedersi riconosciuto questo status in un tempo accettabile, tempi più certi perché i colpevoli siano condannati con maggiore rapidità, come la società siamo allora orgogliosi di fare questa legge; siete voi gli incoerenti. Le vostre proposte più avanzate le avete messe in un cassetto, ma sono stampate. La vostra ipocrisia è palese, anche nei confronti della Corte costituzionale, svillaneggiata da chi a Milano non ha tenuto conto di quella sentenza. Quindi, una legge per tutti cittadini. Noi vorremmo arrivare al giorno in cui ogni cittadino, indipendentemente dal suo cognome e dal suo ruolo in queste istituzioni, venga giudicato con imparzialità dalla magistratura italiana. Temiamo che questo oggi ancora non accada. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP)*. Voteremo convinti questa legge, come abbiamo votato le norme antimafia, come voteremo la riforma del processo penale, come abbiamo votato la riforma del processo civile, come ci occuperemo di intercettazioni, di sicurezza e di tutte le materie importanti. Cari colleghi, richiamando alla memoria la vostra ipocrisia la vostra incoerenza - lo diciamo in conclusione - la legge è contro la irragionevole durata dei processi, perché tempi da 10 a 15 anni sfido chiunque a dimostrare che siano brevi.

Grazie, Presidente. ai colleghi della maggioranza, cui sono legato da amicizia e vicinanza politica, che non metto certamente in dubbio. La devo al presidente Gasparri e al vice presidente Quagliariello, che sono stati anche molto pazienti nella interlocuzione con me su tale questione. La devo al presidente del Consiglio Berlusconi, cui devo la mia candidatura e, stante la legge elettorale, di fatto la mia presenza qui. Voglio anche che sia evitata ogni possibile strumentalizzazione. Credo molto francamente che la maggioranza abbia fatto un errore grave, che è quello di non ammettere pubblicamente che c'erano due obiettivi: quello, condiviso da tutti qui dentro, della ragionevole, certa e breve durata dei processi, e quello, che è diventato una specie di agenda nascosta, della tutela del presidente Berlusconi

Grazie, Presidente. Credo però che l'opposizione abbia fatto l'errore di non ammettere che la tutela del Presidente del Consiglio e dell'Esecutivo dalle persecuzioni della magistratura non è un problema solo di questo Presidente del Consiglio, ma del Paese, atteso che tre delle ultime cinque legislature si sono concluse anticipatamente per via giudiziaria. Credo anche che non abbia ammesso che la lunghezza eccessiva dei processi

Signor Presidente, poiché ho rilevato dall'intervento del presidente Gasparri che lui trova difficoltà a comprendere ciò che in maniera così chiara è stato detto dalla senatrice Finocchiaro, mi limito soltanto ad aggiungere di riflettere bene, perché nel disegno di legge che ci contesta non era presente la retroattività. E chiudo. A più riprese, in Commissione e in Aula, abbiamo tentato, con tutti gli strumenti che la legge ci offre, di

Per queste ragioni e per tutte quelle che abbiamo espresso in questi giorni intendo prendere, in difformità dal mio Gruppo, le distanze, anche fisiche, e dunque mi allontanerò dall'Aula nel momento in cui voi